Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi nel pomeriggio di giovedì 1° settembre, ha approvato il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 15 settembre 2011. La discussione in Assemblea del decreto-legge recante norme in materia di stabilizzazione finanziaria e sviluppo avrà inizio a partire dalla seduta pomeridiana di domani, alle ore 16,30. Come già comunicato ai Gruppi per le vie brevi gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 19 di oggi. Si ricorda che, trattandosi di un provvedimento considerato dal Governo "correlato" alla manovra di finanza pubblica, gli emendamenti privi di copertura finanziaria - come già avvenuto in Commissione - saranno dichiarati inammissibili sulla base del parere della Commissione bilancio. Per la discussione del decreto-legge il calendario prevede un ampio dibattito con sedute ad orario prolungato che si protrarranno, se necessario, fino alla giornata di sabato 10 settembre, per complessive 29 ore di lavoro, delle quali 20 ripartite tra i Gruppi, escluse le dichiarazioni di voto finali. Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 8 settembre, alle ore 10, per procedere alla votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale e di un componente del Consiglio superiore della magistratura. Conseguentemente la seduta antimeridiana dell'Assemblea avrà inizio alle ore 11. La prossima settimana saranno esaminati i seguenti provvedimenti: contributi a enti di ricerca sul Medioevo; professioni sanitarie; attività venatoria in ambiti diversi da quello di appartenenza, nonché il Rendiconto e l'Assestamento del bilancio dello Stato.

vorrei comunicare all'Aula che ho avuto modo di apprendere, da alcuni dispacci d'agenzia dei quali do lettura, alcune significative dichiarazioni dei Capigruppo del Partito Democratico e del La presidente Finocchiaro ha dichiarato: «Siamo pronti a votare la manovra fin da domani pomeriggio, anche in seduta notturna, per concludere i lavori mercoledì. Abbiamo rinunciato agli interventi in discussione generale e notevolmente ridotto il numero degli emendamenti, perché riteniamo importante che la manovra venga discussa e approvata seguendo il normale *iter* parlamentare. Peraltro l'approvazione della manovra mercoledì rende del tutto inutile l'ipotetica apposizione della questione di fiducia, che non risulterebbe giustificata dalla necessità di anticipare i termini dell'approvazione». ha auspicato fin dall'inizio del confronto parlamentare la rapidità dei tempi evitando il ricorso alla fiducia. Lo abbiamo ribadito più volte in questi giorni. Il dibattito in Commissione bilancio ci ha visto aperti ad accogliere, nel rispetto dei saldi, proposte delle minoranze. Con la *spending review* e la norma del condono 2002 abbiamo rafforzato la manovra. Rinunciando ad emendamenti in Aula, siamo impegnati al varo del decreto già nelle prossime ore.

non passeranno venti giorni che il Governo ci presenterà un'altra manovra correttiva (mi pare infatti che si vada in questa direzione), abbiamo la necessità di chiedere al Governo e alla maggioranza di migliorare adesso la manovra, e non tra 15 giorni. Ecco perché, signor Presidente, noi la invitiamo, con fermezza, ad evitare strozzature dei tempi. Se poi il Governo dovesse ritenere di mettere la fiducia, lo faccia, assumendosene la responsabilità: il Paese non si aspetta altro da questo Governo. Pertanto, se vuole andare avanti con il voto di fiducia, lo faccia. Noi riteniamo che ci siano i tempi

grande attenzione a questa fase e ha molta preoccupazione per la condizione del nostro Paese e per la vastità e la profondità della crisi che sta attraversando tutto il mondo occidentale. Assieme alle altre opposizioni

chiesto che questa manovra potesse essere invece discussa in Commissione, ed è stato fatto: alcuni nostri emendamenti sono stati anche accolti. Ciononostante consideriamo la manovra ancora assolutamente inadeguata rispetto alle necessità, e crediamo che una

mia sorpresa per queste dichiarazioni. Ritengo che i tempi siano importanti, ma che il merito sia altrettanto importante: e questa manovra ha bisogno di essere corretta radicalmente, nelle prossime ore,

Siamo molto soddisfatti del lavoro proficuo svolto in Commissione, anche in collaborazione con le opposizioni. Sappiamo bene che il momento impone all'Italia decisioni drastiche, complesse e difficili.